L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dal dott. Luca ZAIA dalla carica di Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali ed ha nominato Ministro del medesimo Dicastero il dott. Giancarlo GALAN. Credo di interpretare i sentimenti di tutti, al di là della diversità dei ruoli, nell'augurare buon lavoro al nuovo Ministro e a tutti i Presidenti di Regione eletti. la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 aprile prossimo. L'ordine del giorno di oggi pomeriggio è integrato con 1'esame del disegno di legge recante sanatoria degli effetti del decreto-legge in materia elettorale non convertito. Per la discussione i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi al fine di assicurare il voto finale - con la presenza del numero legale - entro questa sera. Domani mattina, alle ore 9,30, il Ministro della giustizia interverrà nel dibattito sul disegno di legge di riforma della professione forense. Proseguirà poi la discussione generale, con le successive repliche del relatore e degli altri rappresentanti del Governo. Il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti sul provvedimento è stato fissato per le ore 13 di venerdì 23 aprile, cosicché la votazione sui medesimi possa avere inizio a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 27 aprile. Nella giornata di domani saranno inoltre esaminati disegni di legge di ratifica conclusi dalla Commissione competente e documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Nella mattina di giovedì 22 aprile l'Assemblea non terrà seduta in relazione ad un rilevante impegno politico del Gruppo PdL. Nella seduta pomeridiana dello stesso giovedì 22 avrà luogo, con trasmissione diretta televisiva della durata di un'ora, un'informativa del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanardi sul Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. I rappresentanti dei Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno. Il calendario della prossima settimana prevede, oltre al seguito della discussione del disegno di legge di riforma della professione forense, la mozione Vimercati sull'aeroporto di Malpensa e ratifiche di accordi internazionali. Nel pomeriggio di giovedì 29 aprile, alle ore 16, si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata al Ministro per le pari opportunità, con trasmissione diretta televisiva. La Presidenza ricorderà le figure degli ex senatori Roberto Ruffilli, assassinato ventidue anni fa dalle Brigate Rosse, e Maria Paola Colombo Svevo, deceduta ieri, rispettivamente in apertura della seduta pomeridiana di domani e della seduta pomeridiana di martedì 27 aprile. In entrambi i casi seguiranno gli interventi dei rappresentanti dei Gruppi per 5 minuti ciascuno. Infine, i Capigruppo hanno convenuto sulla calendarizzazione, a decorrere dalla seduta pomeridiana di martedì 4 maggio,

Vorrei esprimere, da parte del mio Gruppo, la vicinanza e i sentimenti di più profondo cordoglio alle famiglie. Vorrei però anche ricordare a tutti noi che nell'isola di Ventotene erano avvenuti altri crolli

chiedeva un intervento sull'isola di Ventotene. Nell'interrogazione chiedevamo esattamente questo: «quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di realizzare un piano straordinario di interventi strutturali per la messa in sicurezza dell'isola di Ventotene con lo scopo di scongiurare seri pericoli per l'incolumità degli abitanti». Il problema della fragilità delle nostre coste e delle nostre isole è molto delicato.

il Governo ritenga che siano soltanto di natura politica. Crediamo di poter stare vicino ai territori segnalando le loro necessità e le difficoltà, soprattutto per le isole minori,

la nostra vicinanza alle famiglie. Ma - ripeto - dobbiamo essere consapevoli che di fronte a simili tragedie ci può essere soltanto un sentimento di dolore, e non ci sono parole in grado

Sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto comprensivo statale di Saonara, in provincia di Padova, ai quali rivolgiamo il nostro saluto e l'augurio per la loro attività di studio per il corrente anno scolastico, che si avvicina alla conclusione.

Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea è stato approvato dalla Camera dei deputati il 15 aprile scorso ed è stato esaminato questo pomeriggio dalla Commissione affari costituzionali. Esso contiene esclusivamente una disposizione di sanatoria degli effetti del decreto-legge n. 29 del 2010, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, emanato il 5 marzo 2010. Come è noto, il 13 aprile il decreto-legge è stato sostanzialmente respinto a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea della Camera, di un emendamento soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. In conseguenza della mancata conversione del decreto, la norma del disegno di legge prevede che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e che siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito. Tale soluzione si rende necessaria poiché le disposizioni del suddetto decreto hanno trovato applicazione in occasione delle recenti elezioni del 28 e 29 marzo in diverse Regioni la Lombardia, la Liguria, il Lazio, il Piemonte, nonché l'Abruzzo e la Calabria per quanto riguarda le elezioni amministrative), fornendo la cornice giuridica affinché la magistratura, sia ordinaria che amministrativa, potesse pronunciarsi senza dubbi ed incertezze su una materia delicata per i diritti dei cittadini, chiamati a rinnovare gli organi rappresentativi regionali e locali. Occorre ricordare peraltro che, oltre al Consiglio di Stato e alla Corte costituzionale, differenti organi giurisdizionali hanno adottato decisioni in materia, facendo riferimento puntuale ai contenuti del provvedimento. In conformità con quanto avvenuto in precedenti occasioni, si rende dunque necessaria una disposizione legislativa che, entrando in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, salvaguardi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto. Ricordo in proposito un precedente del 1995, quando fu adottato dal Governo Dini un provvedimento d'urgenza che prorogava i termini per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni amministrative indette per il 23 aprile di quello stesso anno. Il decreto-legge, in quell'occasione, non fu convertito perché fu sostenuta, da parte dello stesso relatore, la carenza dei presupposti costituzionali, assumendo che non si potessero modificare le regole di una competizione elettorale già aperta. Dopo pochi giorni dalla mancata conversione del decreto, fu approvata una legge (la legge n. 102 del 1995) che sanò gli effetti che nel frattempo quel decreto aveva prodotto. Resta ovviamente inteso che la salvaguardia degli effetti del decreto-legge n. 29 del 2010, così sancita dal provvedimento in esame, riguarda esclusivamente atti e provvedimenti già adottati e rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto stesso, quindi esclusivamente in riferimento alle elezioni che si sono svolte il 28 e 29 marzo e ai relativi ballottaggi. Presso la Commissione affari costituzionali della Camera, ove ha avuto inizio l'*iter* del disegno di legge, come pure in Assemblea, tutti i Gruppi parlamentari, ad esclusione del Gruppo dell'Italia dei Valori, hanno votato a favore del provvedimento. Come emerge dal dibattito, i senatori dell'opposizione hanno ribadito la propria contrarietà al contenuto del decreto-legge, richiamando rilievi e valutazioni già espressi in diverse occasioni. Purtuttavia, si è convenuto sulla necessità di fornire una chiara base giuridica a rapporti e situazioni che si erano ormai prodotti alla luce della normativa del decreto non convertito. Ritengo pertanto auspicabile, in questa sede, che si convenga sull'opportunità di non riaprire la discussione sul merito del decreto non convertito, concordando sulla necessità di concludere l'*iter* normativo aperto con le note vicende che hanno coinvolto alcune liste elettorali in determinate Regioni.

Signor Presidente, colleghi, il provvedimento presente intende sanare gli effetti del decreto-legge n. 29 del 2010, respinto dalla Camera dei deputati il 13 aprile 2010. Il decreto-legge n. 29 presentava profili assai rilevanti di incompatibilità con il dettato costituzionale, in particolare in riferimento all'articolo 72,

la si può intendere pienamente confluibile e trasposta *in toto* agli effetti prodotti dai rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge decaduto e salvati dal presente provvedimento sanatorio. Il vizio costituzionale contagerebbe inevitabilmente la presente normativa. È anche essenziale ricordare che la Corte costituzionale, se dovesse pronunciarsi sul presente provvedimento di sanatoria, potrebbe dichiararne l'incostituzionalità per gli effetti prodotti e i rapporti giuridici nati sulla base di un provvedimento incostituzionale vissuto nell'ordinamento giuridico per 60 giorni e sul quale si è fondata, di fatto, la legittimità ordinamentale delle ultime elezioni regionali. È vero

ma gli effetti giuridici già sorti continueranno a produrre i loro effetti *pro futuro*, se il presente provvedimento sanatorio dovesse essere approvato.

laddove l'articolo 72, comma 4 della Costituzione sancisce invece che: "La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale

in base al quale il Governo non può mediante decreto-legge "provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 2, della Costituzione". Pur avendo la giurisprudenza costituzionale delimitato la materia elettorale cui applicare il divieto di intervento della legislazione di urgenza al "voto" e al "procedimento" elettorale in senso proprio (sentenza n. 161/1995),

e il limite della materia elettorale appare legato ad una motivazione costituzionale che investe direttamente la natura instabile e provvisoria dei decreti-legge e delle caratteristiche del suo procedimento di conversione. un intervento sulla normativa elettorale con questo strumento appare in sé rischioso, se solo si considera che la eventuale mancata conversione del decreto-legge, e la conseguente decadenza dei suoi contenuti normativi, potrebbe avere ricadute pesantissime sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sulla loro validità. Questo punto è stato anche segnalato con precisione dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati organo tecnico a composizione paritaria tra maggioranza ed opposizione - nel parere sul decreto-legge n. 29 del 2010 reso alla Commissione Affari Costituzionali, aveva affermato che: «sul piano dei limiti di contenuto dei decreti-legge, il provvedimento in esame presenta profili problematici, in quanto reca, all'articolo 1, norme in materia elettorale in difformità con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge n. 400 del 1988, secondo Il decreto-legge n. 29 del 2010 non si limita affatto ad essere interpretativo, ma apporta invece vere e proprie innovazioni alla normativa vigente. La pretesa interpretazione autentica recata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 29 era peraltro finalizzata a risolvere problematiche connesse alla reiezione di alcune ben individuate liste elettorali e non invece finalizzata a comporre un contrasto giurisprudenziale, che in occasione delle elezioni regionali del 2010 non si è invece mai realizzato. Per far ciò, il decreto n. 29 si è incautamente addentrato nello specifico (peraltro senza ottenere alcun risultato sul piano giurisdizionale). L'articolo 9, comma 1, della legge n. 108 del 1968 afferma che le liste dei candidati «devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente a quelli della votazione». Pertanto, ciò che deve compiersi nella fascia oraria indicata è la presentazione delle liste, e con tale espressione non si può intendere la «presenza dei delegati nei locali del tribunale», come vorrebbe il decreto interpretativo: ciò, infatti, non sarebbe un significato che l'articolo 9, comma 1, della legge n. 108 del 1968 potrebbe esprimere potenzialmente in virtù di un'interpretazione, ma è una vera e propria integrazione della disciplina del 1968. Quindi, la prima violazione riguarda l'articolo 72, quarto comma, della Costituzione. La seconda, altrettanto grave (e forse anche di più), riguarda l'articolo 122, in cui si prevede: «Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione» - non con provvedimenti interpretativi «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi» e, soprattutto, la violazione della competenza legislativa regionale in base all'articolo 117

la disciplina dell'organizzazione di governo delle Regioni è stata profondamente innovata. Spetta ora ai nuovi statuti, approvati con legge regionale, determinare, in armonia con la Costituzione, la forma di governo delle Regioni e i principi fondamentali della loro organizzazione e del loro funzionamento (nuovo articolo 123, primo comma, della Costituzione). Spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione

Dalla citata sentenza emerge un richiamo alla sentenza n. 376 del 2002 e alla ordinanza n. 383 del 2002 in forza del quale la Corte costituzionale afferma che a "seguito di tale riforma, le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità,

delle sentenze della Corte costituzionale che siamo di fronte ad una precisa violazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

- e sicuramente è così - il presente provvedimento sanatorio. Pertanto, ciò visto, il Gruppo dell'Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, propone di non passare all'esame dell'Atto Senato n. 2111.

nelle questioni che sono state oggetto di tanta discussione al momento del contendere sul decreto-legge

ultroneo richiamarle. In fondo, il senatore Pardi fa dipendere da un'asserita incostituzionalità di quel decreto-legge anche la non costituzionalità del

la Costituzione, senza particolari interpretazioni, vediamo come all'articolo 77, ultimo comma, sia scritto che: «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». Il legislatore costituzionale, in sede di Assemblea costituente, si fece intelligentemente carico della sorte dei decreti non convertiti e stabilì, in una norma di carattere costituzionale, lo ripeto - possono essere regolati con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Credo che poco sia più chiaro di questo So che parte della dottrina è entrata nel concetto dei rapporti giuridici per dire bianco, grigio e nero, ma la la Costituzione deve essere interpretata prima di tutto secondo l'incisività del testo

semplicità: «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29».

della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale»: ciò significa che non si possono approvare leggi elettorali attraverso la procedura legislativa

Intanto, l'espressione contenuta in quella norma non è così chiara come si vorrebbe dedurre, ma sappiamo anche che, trattandosi di una legge ordinaria,

che il provvedimento di validazione e di sanatoria del quale ci stiamo occupando venga in qualche modo messo in forse da quanto è accaduto nella fase precedente. Se interpretiamo correttamente l'articolo 77 della Costituzione e la possibilità di mettere in essere una norma che vada a salvare dei rapporti, ci rendiamo conto di come oggi non vi sia spazio per le obiezioni meditate e ben esposte dal senatore Pardi. D'altronde, come faceva presente il

confermò la possibilità e la conformità al sistema di un tipo di legge come quella che andiamo ad approvare.

Chiedo pertanto che la questione pregiudiziale QP1 venga respinta. Signor Presidente, colleghi, ascoltando con il consueto rispetto e con la dovuta attenzione il senatore Boscetto, mi è venuto in mente quel modo di dire che si usa dalle mie parti, in Sicilia,

il disegno di legge all'esame del Senato è altra cosa: si tratta di un disegno di legge che si limita a regolare i rapporti intervenuti in vigenza del decreto-legge nulla decide ovviamente per il futuro. Per questa semplice ragione, per tutelare l'interesse dei cittadini e in qualche misura delle autorità che hanno applicato quel decreto-legge mentre era in vigore, credo che la questione pregiudiziale non abbia alcun fondamento ed è la ragione per la quale ribadisco

che vi sono degli effetti giuridici già sorti e, dall'altra, che una Regione ha impugnato il decreto-legge del Governo che interpretava le leggi elettorali. Ebbene, quella Regione è la Regione Lazio.

io penso che nell'esaminare questo provvedimento dobbiamo anzitutto farci una domanda rispetto all'atteggiamento da assumere, una domanda che ci possiamo spesso porre, ma in particolar modo di fronte a provvedimenti di questo tipo: cioè, se noi agiamo secondo l'etica della convinzione e, quindi, se noi confrontiamo i nostri principi di partenza con il testo o se, invece, ragioniamo, sempre per restare nella dicotomia di Max Weber, sulla base dell'etica della responsabilità, e quindi ci poniamo il problema di confrontare i nostri principi rispetto al testo, ma con sguardo mirato alle conseguenze che noi provochiamo con un atteggiamento o con un altro sul testo. Infatti, partire dall'etica della convinzione produce delle conseguenze, mentre partire dall'etica della responsabilità ne produce altre, che vado rapidamente a illustrare in quattro brevi punti. primo punto è che noi continuiamo a ritenere la scelta del decreto-legge una grave forzatura istituzionale. Il decreto-legge, per fortuna, è stato respinto alla Camera il 13 aprile, ma vogliamo ricordare che in particolar modo i commi 1 e 4 dell'articolo 1 del decreto presentavano numerosi profili di illegittimità costituzionale, a cominciare dall'idea che essi fossero meramente interpretativi. I commi 1 e 4 erano quelli mirati a salvare la lista del PdL in provincia di Roma. Ora, per cercare di dimostrare la tesi della natura interpretativa di quelle norme, il collega deputato Calderisi, relatore alla Camera, è riuscito a trovare solo una circolare del Ministero dell'interno che impone agli uffici elettorali di ricevere comunque le liste, anche quelle che appaiono irregolari o presentate tardivamente. Il medesimo Calderisi ammetteva, però, che tale circolare, che faceva seguito ad altre analoghe, era costruita per cause di ritardo di forza maggiore e che quelle disposizioni sono state interpretate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato a salvaguardia delle liste solo in presenza di un minimo scostamento di orario: cautela niente affatto riprodotta dalla norma che si voleva interpretativa. Rimando per le obiezioni di costituzionalità alla questione pregiudiziale che il collega Gianclaudio Bressa aveva presentato alla Camera per il Gruppo PD e segnalo che anche la Commissione bicamerale per le questioni regionali, nel suo parere, votato ad ampia maggioranza il 16 marzo, aveva segnalato che c'era un problema nel voler applicare un decreto-legge a Regioni che avevano già legiferato con norme proprie, in attuazione della legge costituzionale n. 1 del 1999. Quindi, il decreto era comunque una grave forzatura:

ci consente di fare un'operazione di sanatoria *ex post* per decreti non convertiti, ma ci dà due modalità molto diverse. Può trattarsi infatti di una pura riproduzione delle norme, la cosiddetta sanatoria per riproduzione: prendo una norma di un decreto decaduto e la rimetto per intero in un nuovo provvedimento. Anche questa non avremmo potuto Anche questa non avremmo potuto accettarla dato che gli elementi di forzatura che c'erano nel testo, al di là dello strumento del decreto, erano comunque anche relativi al contenuto e non solo allo strumento. Altra è quella che si chiama sanatoria per cristallizzazione, quella che stiamo facendo oggi. Una sanatoria per cristallizzazione prende le norme del decreto ma le salva solo per il passato; quindi rende impossibile che le norme siano produttive di effetti per il futuro. La norma del decreto era una norma che andava ad interpretare a regime le elezioni e, quindi, avrebbe avuto effetti anche nelle successive elezioni regionali. La norma di mera sanatoria per cristallizzazione che stiamo facendo salva esclusivamente i risultati delle elezioni regionali, già svolte in questa tornata e che, altrimenti, andrebbero ripetute. Quindi, il decreto faceva un grave errore perché cambiava le regole mentre si stava giocando. Ma se noi non facessimo oggi questa sanatoria per cristallizzazione, cambieremmo le norme dopo che si è giocato: norme a cui i cittadini si sono attenuti perché erano vigenti in quel momento, pur se contenenti alcuni vizi. Terzo punto: analogo precedente si era verificato nell'anno 1995 e una risposta positiva ad una sanatoria di cristallizzazione era venuta allora dal relatore, lo scomparso presidente Leopoldo Elia. Leopoldo Elia. Leopoldo Elia, dopo aver contribuito alla bocciatura del decreto, intervenendo in Aula, invece, favorevolmente sulla sanatoria disse che «non è contraddittorio far salvi gli effetti degli atti al fine di rendere immune da ogni possibile obiezione la validità dell'intero procedimento, in modo che da questo episodio così circoscritto non derivino conseguenze negative per una situazione che è certamente tra le più delicate della vita del Paese, vale a dire una vicenda elettorale». Quarto e ultimo punto, a mo' di conclusione: noi non possiamo oggi che ripetere la logica esposta da Leopoldo Elia. Ci facciamo carico, per responsabilità istituzionale e per etica delle responsabilità, delle regole che vigevano al momento delle elezioni regionali e, solo a questo fine, è ammissibile una sanatoria per cristallizzazione. Con questo manteniamo la dura opposizione che abbiamo fatto al decreto e diciamo che, invece, non avremmo accettato una sanatoria che avesse provveduto di qui al futuro.

Le istituzioni della Repubblica si sono rese responsabili di una serie senza precedenti di omissioni e violazioni di obblighi di legge che hanno negato ai cittadini il godimento dei diritti civili costituzionalmente garantiti. Il Ministero dell'interno non ha impartito, alle oltre 200.000 persone cui la legge affida la funzione di autenticare le firme, le disposizioni necessarie per esercitare utilmente il loro potere e dovere di farlo. Comuni, Province, tribunali e procure non hanno predisposto e organizzato un adeguato servizio pubblico di autenticazione. La RAI, violando quanto previsto dalla legge e dal Regolamento della Commissione parlamentare di vigilanza, ha trasmesso le informazioni relative alle procedure elettorali e le modalità per sottoscrivere le liste di candidati solo negli ultimi sei giorni ed in orari di bassissimo ascolto; nelle passate elezioni regionali di marzo 2010, in sei regioni le leggi elettorali sono state novellate a meno di un anno dal voto, nello specifico le seguenti: Calabria,

Vi ricordo che il Consiglio d'Europa ha raccomandato a tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione europea che le leggi elettorali non possono essere modificate nell'anno precedente le votazioni. La Corte europea dei diritti dell'uomo, un anno fa, ha condannato un Paese per modifiche fatte

per rispettare la volontà popolare, ma di quale volontà popolare si possa parlare nelle condizioni in cui ci siamo venuti a trovare e nelle quali si sono svolte le ultime elezioni regionali, è una domanda che resta certamente aperta. Le condizioni, infatti, erano di assoluta illegalità. Abbiamo cercato di documentarlo in ogni modo, anche con atti e ricorsi che sono tutt'oggi in fase di esame. Il «conoscere per deliberare» è sicuramente venuto meno in una campagna elettorale che ha visto la RAI nel completo silenzio. Le pari condizioni di partenza, che dovrebbero essere ovviamente il minimo indispensabile per assicurare

Ceccanti, poco fa, parlava di un decreto che cambiava le norme; noi, invece, di una legge che cristallizza quel cambiamento. Il decreto non interveniva sull'illegalità e non lo fa neppure questa legge.

inizierò invece con una citazione (magari non a livello di quella del senatore Ceccanti, ma spero di sì): citerò il senatore Ceccanti. Egli ha elaborato il suo intervento su due pilastri: da una parte, l'etica della responsabilità e, dall'altra, la sanatoria per cristallizzazione. L'etica della responsabilità è, o almeno dovrebbe essere, una pratica quotidiana, da adottare non esclusivamente quando si entra nelle Aule del Parlamento ma quando si cerca di esercitare i propri diritti civili, politici ed anche elettorali, sia che si tratti di diritti di elettorato passivo che attivo. Benissimo: non esclusivamente in merito alle regionali del 2010, ma almeno dalle più volte citate regionali del 1995, i radicali hanno sempre denunciato, in virtù dell'etica della loro responsabilità di rispetto dello Stato di diritto (lo ricordava poc'anzi la senatrice Poretti), la patente e sistematica violazione, da una parte, delle leggi elettorali in questione, dall'altra, anche di altre norme internazionali su cui mi soffermerò più avanti, e sicuramente anche tutta una serie di gravissime omissioni da parte del Governo relative al rispetto di queste determinate norme. norme. Se questo è allora il contesto, e non mi pare che nessuno abbia voluto smentire (ahinoi, nessuno si è neanche voluto aggiungere in maniera militante a questo tipo di denunce degli ultimi due decenni), se questa è la situazione, non credo si possa oggi proporre il provvedimento in questione come una sanatoria per cristallizzazione, con la speranza cioè che questa sia una sanatoria che cristallizza, con il documento che siamo chiamati a votare oggi, il problema. Anzi, in virtù dell'incertezza quotidiana del diritto in Italia, si andrà a creare un ulteriore capitolo di giurisprudenza, che però verrà utilizzata in futuro, come sono stati malamente citati i decreti del Governo Dini del 1995 ed i loro successivi accoglimenti da parte del Parlamento in quell'occasione. si interveniva durante il gioco e non, come si è fatto in questo caso, dopo il gioco. Bisogna infatti ben dividere le due fasi: da una parte, la presentazione delle liste e, dall'altra, la tenuta del voto. Noi radicali abbiamo iniziato fin da gennaio e denunciare la sistematica mancanza di rispetto dello Stato di diritto e, avendo approntato il dossier elencato nell'ordine del giorno descritto poco fa dalla senatrice Poretti, siamo arrivati al 24 febbraio a presentare un'interpellanza urgente al Governo che rielencava ancora una volta le violazioni e le omissioni e chiedeva una presa di posizione con modifiche legislative durante la fase fondamentale della presentazione delle liste. Il decreto salvaliste prima e gli effetti che questo decreto produceva poi vanno a sanare delle violazioni di legge. Si tratta di violazioni che, come è stato ricordato, hanno portato la Regione Lazio ad impugnare il provvedimento dinanzi alla Corte costituzionale. Ci sarà un successivo passaggio, e ricordo che la Regione Lazio era governata dal centrosinistra; quindi, quasi per un'inerzia dell'etica della responsabilità, tutto il centrosinistra dovrebbe sostenere la richiesta della Regione Lazio dinanzi alla Corte costituzionale:

Infatti, occorre ricordare che la Corte di Strasburgo ha desunto dall'articolo 3 del Protocollo aggiuntivo della CEDU un vero e proprio obbligo positivo dello Stato di attivarsi per risolvere le difficoltà che possono insorgere dall'applicazione della normativa elettorale, almeno nei casi in cui esse siano tali da pregiudicare l'effettività del diritto di elettorato passivo e attivo. Qui sono stati fondamentalmente privilegiati i diritti dell'elettorato passivo. Qualora - ma questo magari lo scopriremo tra un anno - la Corte europea dei diritti dell'uomo, che denuncia quotidianamente la mancanza di Stato di diritto in Italia, dovesse finalmente rivedere gli effetti di questo disegno di legge - che, ahinoi, anche buona parte della minoranza sosterrà avrà magari nel 2015 la decadenza di molti Consigli regionali contro i quali ci si è stracciati le vesti durante la campagna elettorale.

Desidero, preliminarmente, osservare che il provvedimento di urgenza era stato adottato per assicurare nel miglior modo il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010. Un particolare apprezzamento desidero, poi, rivolgere al relatore, senatore Vizzini, per l'attività svolta in Commissione e per la relazione introduttiva ai lavori di questa Assemblea. Mi siano consentite alcune brevi considerazioni sulla necessità di adottare il decreto-legge e sulla pari necessità adesso di salvarne gli effetti. Più volte, nel corso di questa legislatura, abbiamo avuto occasione di argomentare in merito all'ammissibilità dello strumento del decreto-legge in materia elettorale (riconosciuta laddove si tratti, come nel caso di specie, di provvedimenti riguardanti la cosiddetta legislazione elettorale di contorno, cioè disposizioni volte a regolare la competizione elettorale sotto gli aspetti procedurali ed organizzativi). Il decreto-legge adottato non era intervenuto sul procedimento già avviato e non conteneva norme di carattere innovativo. L'iniziativa di urgenza era limitata, infatti, a recare norme di interpretazione autentica di disposizioni già esistenti nell'ordinamento elettorale. Desidero far presente che la legislazione elettorale, soprattutto in questi ultimi anni, è stata molto sensibile ed attenta a favorire ed a facilitare l'esercizio del diritto di voto, come nei recenti casi, ad esempio, degli elettori intrasportabili o di alcune categorie di cittadini residenti, anche temporaneamente, all'estero. Si possono avere idee e valutazioni diverse sull'opportunità di ricorrere o meno all'iniziativa d'urgenza. Tuttavia, senza un tale intervento, necessitato dalla vicinanza della scadenza elettorale, si sarebbe impedito a taluni cittadini di esercitare il diritto di voto secondo i propri convincimenti. In caso contrario, vi sarebbe stato il rischio concreto di una alterazione del consenso. Le disposizioni sono venute incontro all'esigenza di assicurare la piena partecipazione dei differenti schieramenti alle ultime elezioni. Con le norme contenute nel decreto-legge si è, infine, inteso offrire la cornice giuridica affinché la magistratura, sia ordinaria sia amministrativa, potesse pronunciarsi, senza dubbi ed incertezze, in una materia tanto delicata ma anche altrettanto sensibile per i diritti dei cittadini chiamati a rinnovare gli organi regionali e locali interessati dall'ultima consultazione amministrativa. Ricordo che, oltre al Consiglio di Stato e alla Corte costituzionale, in molte Regioni (tra cui Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto) i differenti organi giurisdizionali, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno infatti adottato decisioni nella materia.

infatti, che un migliore rapporto di cooperazione tra soggetti chiamati a svolgere funzioni riconosciute dalla Costituzione possa essere costruito con una legge che eviti la rincorsa davanti agli uffici nei quali si presentano le liste elettorali e stabilisca un modo più disciplinato di cooperazione tra soggetti

a seguito di quei fatti e di quelle valutazioni si era chiesto un impegno al Governo. Evidentemente i fatti che hanno portato a quel decreto non vengono presi in considerazione dal Governo e dal relatore. Ciò nonostante, se c'è un impegno del Governo a rivedere non solo la consegna delle liste,

pregiudiziale del collega Boscetto che ho ascoltato con attenzione. Non è naturalmente questa la sede per fare la replica della replica (me ne guardo bene), ma voglio soltanto osservare che nella sua interessante risposta manca qualsiasi cenno

dal punto di vista polemico, questo aspetto, forse ciò rappresenta una falla nel suo ragionamento, ma è una cosa che verrà accertata in una discussione amichevole. Quanto al merito politico di questa vicenda, mi allontano vigorosamente dalla materia dell'incostituzionalità che ho cercato di trattare in

che sulla vicenda delle mancate liste a Roma si è scatenato un putiferio mediatico di proporzioni scandalose, e questo naturalmente è stato reso possibile dal fatto che, purtroppo, come non smettiamo mai di lamentare, l'intera vita pubblica italiana ormai è stata e continua ad essere inquinata alla radice dallo strapotere sui mezzi di comunicazione che, di piramide in piramide sovrapposta, fa comunque capo al Presidente del Consiglio. Su questa storia delle liste mancate, rifiutate, sabotate nel collegio romano è stato fatto non solo un putiferio terribile, ma sono state anche accumulate una quantità di menzogne che hanno qualcosa di stupefacente. La vicenda è stata presa a pretesto prima per attaccare i colleghi radicali, dicendo

Cari colleghi, c'è stato un gruppo di un partito preciso che si è dimostrato incapace di presentare le liste e poiché è stato incapace, di fatto, gli elettori che avrebbero voluto e potuto in altri termini coronare il loro sogno di voto sono stati impediti da da questo tipo di incapacità, di inettitudine, di trascuratezza, di non so cosa. Questo non viene affermato

che, alle ore 12, l'area in precedenza individuata è stata chiusa e delimitata dal personale delle forze dell'ordine senza che all'interno vi fosse un delegato del PdL, che non è quindi mai stato espulso dalla predetta area (si è anche parlato di espulsione forzosa). dice che solo alle ore 12,30 un delegato del PdL tentava di accedere all'area con in mano una cartellina, ma non veniva ammesso essendo fuori termine (vedi verbale dei carabinieri dice che il contenitore con i documenti per la presentazione della lista del PdL, lasciato incustodito all'interno della predetta area, è stato dapprima rinvenuto e sorvegliato dai carabinieri, poi prelevato da un delegato del PdL e successivamente riconsegnato agli stessi carabinieri alle ore 19,30 circa. Al

lista e la indicazione dei due delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista (verbale di acquisizione dei carabinieri). A tutti questi dati storici si aggiungono altre considerazioni, sempre del Consiglio di Stato, gli elementi di prova forniti dall'appellante possono al più dimostrare la presenza di almeno un delegato nella fase antecedente la scadenza dell'orario prescritto, ma non il possesso dei documenti. Segue un elenco sterminato un elenco sterminato di altre considerazioni storiche da cui estrapolo solo alcuni punti. Il contestato omesso ricevimento da parte dell'ufficio elettorale della documentazione, anche se presentata tardivamente, non assume rilievo, in quanto avrebbe comunque dimostrato il possesso di una determinata documentazione in orario ampiamente successivo ampiamente successivo alle ore 12. Le dichiarazioni rese in diverse date dagli stessi delegati del PdL, oltre a non essere del tutto coerenti tra le varie versioni, non costituiscono comunque elementi di prova attendibili e via dicendo. Le Le successive relazioni di alcuni carabinieri, invocate dall'appellante, dimostrano solo il possesso da parte di un delegato del PdL di una cartellina, sempre al momento del tentativo di accesso ai locali destinati alla presentazione delle liste, ovvero dopo le ore 12,30 in tempo non utile anche ai sensi del decreto-legge n. il primo reclamo, presentato dai delegati della lista PdL alle ore 17 del 27 febbraio e prodotto in giudizio, conferma la non completezza dei documenti.

1, comma 1, del decreto-legge n. 29 del 2010 e richiamate dal comma 4 dello stesso articolo per la presentazione della lista entro il nuovo termine fissato dal decreto-legge, mancando la dimostrazione del possesso in capo ai delegati della «prescritta documentazione» e non potendo essere condivisa la tesi dell'appellante circa la necessità della sola prova della presenza nei locali del tribunale all'orario prescritto. Credo che una lettura collettiva di questo documento illustrerebbe molto meglio di tanti discorsi il processo di falsificazione sistematica che è stato condotto sui principali mezzi di comunicazione a proposito di questa vicenda che si conclude, naturalmente, con una sanatoria. E come poteva essere diversamente? Abbiamo cominciato sanando il falso in bilancio; si continua sanando tutto ciò che è possibile sanare e, quindi, si sanano anche dei provvedimenti incostituzionali per rimediare, come dice argutamente il collega Ceccanti, con una cristallizzazione di tutto questo pasticcio. È evidente che di fronte a questo pasticcio non possiamo che essere contrari, contrari, contrari. Non c'è nessuna razionalità legislativa in questo modo di procedere

contrario. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, a dir la verità il presidente Vizzini è stato abbastanza cauto: si è attenuto al merito di questo provvedimento senza richiamare la natura o senza, in qualche modo, entrare nel merito del provvedimento precedente. Questo forse è anche opportuno perché questo provvedimento è maturato in un contesto che dal punto di vista politico non possiamo ignorare. Questo contesto è stato contrassegnato nella maggioranza di Governo da confusione, scontri interni, incompetenza, improvvisazione, soluzioni pasticciate. Non ha certo dato al Paese un'immagine del saper fare, né del saper ben fare. Non è vero che i cittadini non siano stati turbati da questi passaggi confusionari e anche vagamente destabilizzanti mentre era in corso una competizione elettorale. Le astensioni che hanno colpito in alcune Regioni e in tutto il Paese la coalizione di Governo risentono, anche se in piccola parte, anche del clima che si è determinato su questa vicenda. Un tratto caratteristico ne è stata l'arroganza con cui si è voluto riparare agli errori che erano stati commessi, non volendo tematizzarli e producendo interventi ancor più gravi dal punto di vista politico, istituzionale e giuridico. Mi riferisco al decreto-legge che è stato caducato dalla Camera. Il Capo dello Stato ha mostrato in una situazione già viziata e compromessa, ancora una volta saggezza, sobrietà, senso della responsabilità per dover necessariamente bilanciare e salvaguardare gli interessi costituzionali e di tutti gli italiani. Questa maggioranza ha messo in campo errore su errore: nella presentazione delle liste, nei ricorsi, intervenendo in materia elettorale con decreto-legge, mentre appunto era aperta una procedura elettorale. Questo decreto-legge è stato dal Gruppo del PD fortemente criticato dal punto di vista politico e giuridico. Dal punto di vista politico non si è avuta nemmeno la serietà di chiedere scusa agli elettori italiani degli errori e dei pasticci causati e di richiedere alle forze politiche tutte la possibilità di un provvedimento legislativo, che pur poteva adottarsi, come male minore rispetto alla decretazione di urgenza, che ha rischiato di far scrivere una brutta pagina nella storia delle istituzioni parlamentari. Dal punto di vista giuridico il provvedimento era viziato da incostituzionalità sul piano generale e anche per quanto attiene al riparto delle competenze previste dall'articolo 117, essendo la materia elettorale di competenza regionale per le Regioni che già avevano deliberato in tal senso. Oggi ci sorprende ascoltare ancora, dopo che la Camera a maggioranza ha bocciato il decreto-legge, argomentazioni difensive che richiamano le categorie di legislazione interpretativa, di norme di contorno, come qualcuno le ha definite.

costruivano l'irragionevolezza di una irretroattività, come ha affermato il collega Ceccanti nel suo intervento, a favore di situazioni ben precise e ben identificabili. Il provvedimento odierno ci richiama al senso di responsabilità istituzionale e costituzionale, non solo perché i cittadini hanno votato. Ricordiamo le parole dello stimatissimo, allora relatore, professore Leopoldo Elia, che nel 1995, in un precedente quasi analogo tenne a precisare quanto non sia contraddittorio far salvi gli effetti degli atti al fine di rendere immune da ogni possibile obiezione la validità dell'intero procedimento, in modo che questo episodio sia circoscritto e che da questo non derivino conseguenze negative per una situazione che è tra le più delicate del Paese, cioè la vicenda elettorale. Il provvedimento in esame ci richiama alcuni principi fondamentali dal punto di vista costituzionale e alcune questioni di certa rilevanza: il valore del voto e la sovranità popolare. Non a caso, però, anche il fatto di potere, con legge, regolare quanto previsto da un decreto-legge che non viene convertito. Questo non è di poca influenza. Non a caso i nostri Costituenti, avendo fatto espressa previsione con l'articolo 77 di poter far salvi gli effetti di un decreto-legge non convertito, usano molta prudenza sull'uso del decreto-legge, ma, al tempo stesso, prevedono la possibilità per le Camere di regolare appunto i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti. È in gioco un principio fondamentale al quale ci ispiriamo e crediamo bisogna ispirarsi: quello dell'affidamento e della sua tutela, in virtù del quale i cittadini, che non sono responsabili degli errori prodotti, e l'amministrazione in senso astratto, hanno applicato norme che erano valide. Pertanto, le stesse ragioni che ci hanno portato a opporci al decreto-legge, che ci hanno fatto proporre l'emendamento approvato dalla Camera che ha travolto il decreto-legge, ci impongono di impedire che si venga a determinare una situazione anomala ancora più grave: che il voto popolare che si è espresso possa essere travolto dall'irresponsabilità e dall'incompetenza di chi ha prodotto errori formali e che ha voluto ostinatamente adoperare la strada del decreto-legge. Le istituzioni parlamentari si sono difese. Non avete - voi della maggioranza - eliminato le brutte figure politiche, ma le avete raddoppiate. Voi avete piegato la forza della legge, come spesso siete abituati a fare, per senso particolare e per interessi di parte. Noi abbiamo condotto una battaglia di rispetto per le leggi e per le istituzioni parlamentari. Le ragioni della politica hanno prevalso fortunatamente sui numeri e siamo soddisfatti di questa battaglia, per questo senso di lealtà verso le istituzioni, verso i principi di rispetto della legalità che bilanciano e regolano gli interessi nella nostra Carta costituzionale. Per rispetto della competizione elettorale e del principio dell'affidamento, noi volgiamo il nostro voto non per interessi di parte, ma nell'interesse del Paese ed è per queste ragioni che esso sarà favorevole.

Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà.

un consenso forte, *bipartisan*, che lo sostiene. Si perde decisamente di vista l'interesse generale degli elettori, dei cittadini e degli italiani e si va a privilegiare quello particolare,

Signor Presidente, anch'io voterò contro il disegno di legge in esame. Il relatore Vizzini ha voluto liquidare come ulteriori polemiche le premesse dell'ordine del giorno G100, che non sono state accolte né da lui né dal Governo e anche alcuni elementi emersi dal dibattito. Ebbene, quelle non sono ulteriori polemiche: quelle sono denunce circostanziate, documentate, per le quali nessun membro della maggioranza o del Governo ha trovato cinque minuti di tempo da dedicarvi per cercare di rispondere, magari considerandole sì ulteriori polemiche; questo tipo di giudizio ci viene invece proposto in sede di ratifica parlamentare. Oggi - e non credo che si possa sostenere il fatto che le istituzioni parlamentari si sono salvate, purtroppo - per via parlamentare, si va a scrivere l'ultimo (ma in questo caso è sempre il penultimo) capitolo di quello che i Radicali chiamano, ormai da 20 anni, il «caso Italia», cioè la mancanza di rispetto dello Stato di diritto, la totale incertezza - unica certezza - delle regole e, quindi, il distaccarsi progressivo e continuato dell'Italia dalla pratica della regola democratica. Per tutti questi motivi, anch'io voterò contro

la formula potrebbe sembrare un po' inconsueta, ma francamente non so a quale altro momento parlamentare affidare questa mia mozione di sentimento;

a che cosa c'è di pericoloso riguardo alla mafia. In tale conferenza venivano riconosciuti - ed è qualcosa che riconosciamo tutti

gli importanti risultati ottenuti dai magistrati e dalle forze dell'ordine, in una conferenza stampa ufficiale il Presidente del Consiglio dica che

che tutto ciò sia gravissimo e che il Presidente del Consiglio debba rispondere alla domanda che ha posto Saviano nel suo articolo: «Il potere mafioso è determinato da chi racconta il crimine o da chi commette il crimine?».

Il silenzio è uno strumento che la mafia gradisce, infatti per oltre un secolo i mafiosi hanno fatto dell'omertà un totem intangibile.

non ho aggettivi per rendere chiaro quanto tutto ciò mi sembri un'emergenza - il fatto che il Presidente del Consiglio faccia lo stesso invito che boss mafiosi hanno rivolto a questo giovane scrittore nel processo "Spartacus". Signor